L'ordine del giorno reca la discussione delle dimissioni presentate dal senatore Nicola Di Girolamo. Ricordo che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la votazione avrà luogo alle ore 12. Ha chiesto di intervenire il senatore Di Girolamo. Ne

ho rassegnato le mie dimissioni dalla carica di senatore della Repubblica italiana. Dopo tanto fango, dopo l'ignominia di un'esposizione mediatica che mi ha descritto agli occhi del Paese come un mostro, usurpatore della politica e del mandato elettorale, credo fermamente che sia arrivato il momento della responsabilità e della verità dei fatti. Sono convinto di dover rendere disponibile la mia persona, la mia storia personale, la mia esperienza recente, perché chi dovrà giudicarmi possa davvero conoscere i contorni di una vicenda che non è tutta criminale e che potrà finalmente essere vagliata lontano dai riflettori e dal clamore delle prime suggestioni. Sono entrato nell'Aula del Senato forte di una delega affidatami da 24.500 elettori di tutti i Paesi europei, 24.500 cittadini italiani né mafiosi, né delinquenti. Di una piccola parte di costoro avrebbe abusato un gruppo di individui probabilmente inquinati da frequentazioni criminali. Non mi interpreti come troppo ingenuo, signora Presidente, non ero consegnato anima e corpo a questi figuri. La frenesia della campagna elettorale mi ha spinto a valutare poco e male, e lei, mi auguro, immaginerà che non si diventa mafioso nello spazio di un mattino, colpevole come sono di uno o due incontri disattenti. Sono entrato in Senato da professionista del diritto incensurato. La mia non è stata una storia semplice. Orfano già in fasce di un prestigioso economista docente universitario, figlio unico, educato al rigore e alle buone maniere da una madre nobile, ho da sempre ho da sempre dovuto provvedere al sostentamento della mia famiglia e sono rimasto negli anni quello che ero: una persona perbene, incapace tuttavia di difendersi innanzi alla protervia dei malevoli e dei menzogneri. In politica ne ho incontrati alcuni, figli di un'altra storia, ben diversa dalla mia, capaci di fagocitarmi nella smania delle promesse. Ho ceduto, certo, signora Presidente, ma le mie colpe verranno circoscritte dalla verità che saprò esporre ai magistrati cui ho deciso di consegnarmi, forte della convinzione di collaborare alla ricerca della verità e della certezza che dovrò riscattare faticosamente il mio onore innanzi alla mia famiglia, ai miei amici ed all'Assemblea del Senato alla quale ho partecipato con orgoglio e dedizione. Intendo con questa ferma decisione allontanare dalla Camera Alta del nostro ordinamento l'ignominia che mi ha riguardato e che saprò ricondurre alle circostanze ed ai fatti che possono essermi ascritti; quelli, signora Presidente, che riguardano le mie responsabilità e non certamente i contorni di un quadro di compromissioni che oggi mi vengono attribuite ma che non appartengono al mio vissuto reale. Le chiedo scusa, signora Presidente, di averle procurato imbarazzo. Le scuse più profonde le devo tuttavia a mia moglie ed ai miei figli per quanto hanno patito in questi giorni terribili. Dovranno fare a meno della mia presenza per un lungo tempo. Sarà durissima per me e per loro, ma avrò guadagnato con questa sofferta decisione l'orgoglio del riscatto per me, per il Senato, per la politica tutta. Forse sarò l'unico ad essere ricordato per aver rassegnato le dimissioni: è un evento davvero poco usuale in questo drammatico momento di storia nazionale. Non importa. Mi affido alla Provvidenza pronto a sfidare ogni falsità, confidando nella verità ed abbracciando con la mia famiglia il progetto di Dio in Cristo, sperando nella vocazione posta nel cuore e nella mente di ogni uomo. Un'altra parola solamente, Presidente. Avevo scritto questo appunto perché volevo che fosse ben chiaro il percorso che ho voluto e che dovrò affrontare. Vorrei solamente dedicare due parole all'Assemblea per dire che è stata per me una esperienza esaltante ed altissima poter far parte di questa Camera Alta. Non ho assolutamente portato all'interno dell'Aula l'indegnità della 'ndrangheta o della mafia, così come mi è stato ascritto. Ho visto una serie di fotografie sui giornali. Vorrei che chi è qui con me in questo momento riflettesse su in campagna elettorale. In quell'evento specifico, quella sera, ho fatto circa 250 fotografie davanti a quella torta. Vi era quel signore, che dicono essere un mafioso, che a me era stato presentato come un ristoratore, proprietario di una catena di ristoranti anche all'estero, quindi persona con relazioni per poter votare all'estero. Ho fatto la fotografia davanti a quella torta successivamente con il parroco del paese, con il sindaco, con il maresciallo dei carabinieri, con 300 persone. Credo che anche voi abbiate fatto delle fotografie e non credo che abbiate preventivamente chiesto in campagna elettorale i documenti o i carichi pendenti alle persone che hanno fatto le fotografie con voi. voi. Però per queste foto, e nel giro di tre giorni, è stata completamente annientata la mia vita, la mia vita professionale, politica e quant'altro. Vorrei in ogni caso ringraziare tutti gli appartenenti al Gruppo con i quali mi sono onorato di condividere questi due anni della mia vita. Non farò dei nomi, Presidente e colleghi, e me ne scuserete, perché qualsiasi nome facessi oggi, visto che io sono l'untore ed il Lucifero della situazione, se mi riferissi ad un collega chiamandolo per nome si direbbe che lo stesso è colluso con me ed è mafioso. So che i colleghi sanno a chi è diretta diretta questa indicazione di amicizia e di riconoscimento, ma per loro stessa tutela non li richiamerò nome per nome. Ciò vale anche per alcuni componenti dell'opposizione che sono stati vicino a me in alcune realtà, in alcuni sogni: il sogno di poter fare qualcosa a livello internazionale, per aiutare l'ingresso della Turchia in Europa, per un riconoscimento di Cipro, per ragioni che sicuramente esulano dalla mia vicenda personale, che sono alte, altissime e che non voglio minimamente infangare.

parte di un circuito virtuoso e, quindi, un'opportunità e non un problema come da sempre sono stati considerati. Pertanto, con tutte le modifiche che riterrete opportuno apportare a talune modalità

- se lo consente - sarà dedicato anche ad una questione relativa all'ordine dei lavori e ad un richiamo al Regolamento, su cui spero e mi auguro che la Presidenza possa fornire una risposta.

e dalla maggioranza di votare secondo questo ordine: ne prendiamo atto, non la condividiamo, ma la rispettiamo come ogni decisione assunta in quest'Aula. Con analogo senso di rispetto,

e cercando - anche per dare all'Assemblea un senso di serietà e di decoro - di evitare polemiche sterili e strumentali che in questi momenti non hanno alcun significato e peraltro non appartengono alla nostra storia storia e alla nostra tradizione. Dunque, prendiamo atto ed apprezziamo il gesto del collega Di Girolamo; rispettiamo la sua scelta, anche quella di difendersi dalle accuse che gli sono state mosse senza utilizzare o abusare della sua funzione.

Non vogliamo essere iscritti al partito degli ipocriti e dei sepolcri imbiancati e riteniamo giusto che ciascuno si assuma le proprie responsabilità, come ha fatto il collega Di Girolamo in questa circostanza. Detto questo, signora Presidente, ho il dovere di sollevare due questioni. La prima riguarda i nostri lavori a seguito dell'eventuale accoglimento delle dimissioni da parte dell'Aula. Se è infatti vero che l'accoglimento delle dimissioni del collega Di Girolamo da parte dell'Assemblea produce come effetto naturale e regolamentare la preclusione delle mozioni nella parte in cui queste

della mia mozione, che non ha proposto la decadenza del collega Di Girolamo ma la revoca dell'ordine del giorno De Gregorio approvato

delle mozioni presentate dai colleghi Malan e Sanna, nella parte in cui chiedono chiedono la revoca di quell'ordine del giorno. Salvo che, signora Presidente, non vi sia una soluzione che la Presidenza ritenga più funzionale a far sì che quella deliberazione dell'Aula non sia considerata precedente e non faccia stato per il futuro. Anche perché il Presidente del Senato, cito testualmente,

ha chiesto che la Giunta non tenesse conto, nel riesaminare la questione relativa alla decadenza del collega Di Girolamo,

chiesto che quella deliberazione non fosse considerata precedente ai fini del riesame di questa vicenda. Com'è noto, la Giunta, giustamente, ha dovuto precisare al Presidente del Senato che quella decisione poteva essere riesaminata e revocata solo dall'organo che l'aveva posta in essere, e cioè l'Assemblea, e quindi ha dovuto, suo malgrado, prendere atto che quella decisione ha la dignità di precedente cui gli organi di giustizia interna del Senato devono uniformarsi.

reputa opportuno che sull'ordine del giorno presentato dal senatore De Gregorio e approvato dall'Aula

chiedono la revoca di quella deliberazione, è evidente che i Gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione ritengono che quella deliberazione costituisca precedente e quindi un vincolo rispetto alle future decisioni che la Giunta delle elezioni e l'Aula debbano in casi simili o identici assumere. E poiché, signora Presidente, noi leggiamo dai giornali che analogo o simile problema potrebbe verificarsi con riferimento al subentro del dottor Fantetti, che sembra essere dipendente a contratto del Ministero delle politiche comunitarie da prima della elezione, e uno dei requisiti - da quel che mi risulta, ma non vorrei sbagliarmi, però lo pongo in termini problematici e costruttivi e costruttivi - per poter assumere lo *status* di pubblico impiegato è la residenza nel Paese nel quale si presta la propria attività lavorativa (segnatamente nel Comune di Roma) è evidente che questa è una circostanza che la Giunta delle elezioni dovrà in qualche modo apprezzare. Qualora questo apprezzamento fosse espresso non solo da parte della Giunta (il che sarebbe fisiologico) ma anche, eventualmente, da parte dell'autorità giudiziaria (il che sarebbe patologico), è chiaro che varrebbe il principio fissato nell'ordine del giorno De Gregorio e cioè che fino a quando l'eventuale indagine della magistratura non si concluda

opportuno, al di là della questione procedurale, che l'Aula, all'esito del voto sulle dimissioni del collega Di Girolamo, si pronunci sulla mozione da me presentata e sulle parti delle mozioni presentate dai colleghi di maggioranza ed opposizione che attengono specificatamente a questo tema.

L'altra questione estremamente importante è che l'effetto del voto sulle dimissioni del collega Di Girolamo pone una questione relativa alla interpretazione e all'applicazione delle regole sul subentro. A seguito della entrata in vigore della legge Calderoli

e questa convenne - che, fatta eccezione per i casi specifici della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, espressamente previsti dallo Statuto di quelle il procedimento per l'attribuzione dei seggi che si rendano vaganti nel corso della legislatura è un procedimento complesso, che si svolge attraverso fasi diverse e coinvolge le competenze di una pluralità di organi; l'ufficio elettorale regionale, nel proclamare i candidati eletti, consacra l'ordine dei candidati che seguono in ciascuna lista elettorale; che, quando si verifichi la vacanza, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari prende atto dei candidati subentranti ai senatori cessati dal mandato parlamentare e ne dà comunicazione al Presidente; sulla base delle comunicazioni della Giunta, il Presidente del Senato proclama senatori i candidati individuati mediante tale procedura e ne dà comunicazione all'Assemblea, che ne prende atto. Come si vede, la lacuna fu colmata solo per il caso delle elezioni nazionali, visto che per la circoscrizione Estero nulla si dice, pur essendo questa già esistente ed essendo in quella data già presenti in Senato alcuni senatori in essa eletti. Potrà apparire sgradevole, ma è giusto che ricordi che, ad esempio, in quel momento era pendente il ricorso elettorale della collega Giai contro il senatore Pollastri per un errore nei conteggi ammesso dallo stesso presidente dell'ufficio centrale della corte d'appello nell'audizione in Senato del 14 novembre 2006. Incidentalmente, vorrei dire che sono lieto che oggi il senatore Berselli abbia presentato al riguardo una proposta di riforma del voto all'estero, anche se ci saremmo aspettati che, nel caso della collega Giai, essendo lui componente della Giunta, accelerasse i tempi e vedesse in qualche modo garantito il diritto della collega a subentrare allora in Parlamento e non grazie agli elettori in questa legislatura. Comunque, dal punto di vista regolamentare, signora Presidente, il parere del presidente Marini è inapplicabile alla circoscrizione Estero. Lo stesso criterio individuato nel parere diverge da quello previsto dall'articolo 16 della cosiddetta legge Tremaglia. Vi è quindi un'altra ragione di natura regolamentare. Concludo, per non aggravare la sua insofferenza e quella del collega che parlava al telefono prima e che stavamo disturbando. È chiaro che tutto questo comporta un problema, cosa dovrà fare la Giunta per le elezioni dopo le ore 12, in sede di individuazione del subentrante al collega Di Girolamo: della lista così come è stata individuata o se debba - come è possibile che avvenga, considerato che questa normativa e anche i precedenti non si applicano alla elezione nella circoscrizione Estero - iniziare subito una verifica

per la serenità del Senato, devono essere comunque oggetto di un esame e di una valutazione. Chiedo pertanto la cortesia, signora Presidente (senza voler disturbare troppo, ma credo sia una questione istituzionalmente molto delicata, visto che fino ad oggi questa procedura è stata, per volontà di tanti, certamente non nostra, pasticciata), di volerci dare una garbata, cortese ed efficace risposta.

preannunciare che dopo la votazione delle dimissioni, ove le stesse siano accolte, riproporremo il richiamo al Regolamento che ha fatto il senatore D'Alia.

devo riconoscere che sento un certo disagio a svolgere questo intervento. È dal 2006 che si parla dei brogli elettorali nella circoscrizione Estero, inquinando l'immagine degli italiani all'estero, dimenticando in realtà che i veri problemi sull'esercizio del voto all'estero hanno radici in Italia, nella mala-politica italiana e nella criminalità italiana. Le operazioni vergognose che si sono fatte all'estero hanno sempre un'origine in Italia e ben poco hanno a che vedere con gli italiani all'estero. il signor Di Girolamo ha detto una cosa giusta: ha avuto 24.000 preferenze e sicuramente moltissimi di quei voti sono di cittadini italiani residenti di cultura di centrodestra, che hanno votato un candidato del centrodestra; è del tutto legittimo, non vedo cosa vi sia di strano, anche se lui non è residente all'estero. È difficile su un collegio grande come un continente conoscere tutti i candidati.

brogli! Questo non è un problema di destra o di sinistra. Credo che i miei amici emigrati che appartengono idealmente all'altro schieramento siano stati ingannati, siano vittime della truffa che è stata compiuta sulla candidatura del signor Di Girolamo. Non mi pronuncio sui fatti di oggi: per questo, la magistratura farà il suo lavoro.

È a questa domanda che dobbiamo rispondere, ma finora la risposta alla stessa non è stata rassicurante da tutte le parti politiche, perché i problemi delle candidature che emergono oggi nel centrodestra fanno capire che non è stata presa molto sul serio questa circoscrizione; ma per chiarezza ed onestà voglio dire che anche nel mio partito non è stata presa molto sul serio. So che attualmente è un funzionario il responsabile del mio dipartimento, dunque non vedo una grande lettura politica della nostra presenza in questo Parlamento. Credo sia questa la domanda alla quale dobbiamo rispondere. Sono convinto dall'inizio che la presenza dei parlamentari all'estero in questo Parlamento importante per l'Italia più che per gli italiani all'estero; è importante per l'immagine dell'Italia nel mondo, perché l'immagine vera dell'Italia nel mondo non è quella che ci raccontiamo.

Contro questa immagine ci sono milioni di italiani che tutti i giorni lavorano e si impegnano socialmente e politicamente. Ha ricordato in questi giorni l'onorevole Tremaglia che ci sono quasi 400 parlamentari d'origine italiana in tutti i Parlamenti del mondo. Queste persone salvano e ripuliscono l'immagine dell'Italia nel mondo. Per questo motivo è importante la presenza in questo Parlamento, per la promozione del Paese e per portare anche un'altra cultura politica, che non è sempre all'altezza della retorica che sento qui perché noi siamo piuttosto abituati ad affrontare i problemi, a parlare dei problemi concreti ed a cercare soluzioni, accordi ed intese. Questa è la motivazione della nostra presenza e a questo dobbiamo dare una risposta. L'onorevole Tremaglia si è impegnato una vita per ottenere questo voto e noi siamo riconoscenti; però egli non ha ascoltato le nostre proposte quando si è fatta la legge di applicazione sul voto all'estero. In quegli anni nel Consiglio generale degli italiani all'estero abbiamo presentato proposte per il sistema di voto all'estero che si basavano sull'esperienza di altri Paesi che utilizzano il voto per corrispondenza da anni, da decenni. Noi abbiamo voluto inventare un sistema italiano: questo sistema non funziona.

a proporre la riforma della legge sul voto all'estero. Ringrazio il presidente Schifani che, non solo ha autorizzato quell'indagine, ma l'ha disposta in sede congiunta con la Commissione affari costituzionali. Adesso bisogna accelerare questo lavoro, bisogna portarlo fino in fondo per poter fare delle proposte serie di riforma. Questo lo abbiamo chiesto subito dopo il voto, prima che scoppiasse il caso Di Girolamo. Mi avvio a concludere rilevando alcune questioni che mi sembrano abbastanza pesanti per noi. Nella stampa si è letto di tutto, addirittura che il Consiglio generale degli italiani all'estero, tramite un suo membro, il consigliere Ferretti, sia implicato nella vicenda Di Girolamo: questa è un'affermazione gravissima uscita sulla stampa. Il Consiglio generale degli italiani all'estero è un organo consultivo, che nulla ha a che vedere con l'organizzazione e lo svolgimento delle elezioni

sì o no alla presenza dei parlamentari all'estero? Se ritenete che è importante per l'Italia, rispondete sì. Se pensate che è importante per noi all'estero, sono il primo a dire di no: noi ci impegniamo per la nostra integrazione in altri Paesi. Se la risposta è positiva, dobbiamo però essere coerenti coerenti e ciò vuol dire avere rapporti chiari con persone che rappresentano le comunità italiane all'estero. Vuol dire mettere i limiti necessari a tutte le speculazioni che si possono fare sulla nostra pelle. Nascono partiti degli italiani nel mondo; nascono fondazioni per gli italiani nel mondo e sarei felice se il collega De Gregorio potesse spiegare a quest'Aula che tutte le risorse della sua fondazione sono - come spero

di lui non hanno bisogno e di cui non hanno mai chiesto. Gli italiani all'estero hanno bisogno di ben altre cose, hanno bisogno di un'altra politica del Governo nei loro confronti, perché mai come in questi anni siamo stati penalizzati e tartassati.

la politica italiana butta il bambino e mantiene l'acqua sporca: cerchiamo questa volta di non fare la stessa cosa.

non c'è proprio bisogno di essere degli sciacalli o dei maramaldi per inquadrare con onestà, senza ipocrisie, in tutta la sua portata, il fatto gravissimo non tanto della illegittimità, della decadenza e/o delle dimissioni di un senatore della Repubblica, quanto delle cause che hanno determinato una situazione di disagio e danno, forse senza o con pochissimi precedenti per l'immagine, la sensibilità e la dignità di quest'Aula e, di riflesso, dei suoi singoli componenti. Come se non bastasse, il vento furioso dell'antipolitica già soffia in una società delusa che non si sente adeguatamente rispettata e tutelata dalle istituzioni. Infatti, senza pretendere di anticipare le risultanze del prossimo inevitabile percorso giudiziario del caso Di Girolamo, credo si abbia, almeno fino a questa data, per la prima volta un'evidenza netta, circostanziata, più che sufficiente, abbondante, di un intervento diretto, palpabile, comprovato e quantificabile della criminalità organizzata in operazioni di voto politico, approfittando delle smagliature in un sistema elettorale men che ideale, a cui bisogna porre mano subito nella circoscrizione Estero. Intendiamoci. Voglio ricollegarmi all'osservazione del collega Micheloni circa la radice esclusivamente italiana dei mali riscontrati e lamentati all'estero. Non che sia mai mancata, dalle prime elezioni democratiche del secondo dopoguerra ad oggi, un'evidenza spesso aneddotica ma credibile, una percezione forte di pesanti condizionamenti nelle consultazioni popolari da parte della criminalità organizzata in talune realtà locali anche sul territorio nazionale. Tutt'altro. Tuttavia, è capitato per sfortuna, nella prima fase storica dell'esercizio del diritto di voto all'estero, di quella che è stata e resta un'autentica conquista di civiltà e democrazia che altre nazioni europee quali Francia e Grecia ci invidiano, stanno studiando e si preparano ad adottare - ripeto - in questo delicato settore e momento della rappresentanza parlamentare, di toccare con mano uno sciagurato episodio d'inquinamento mafioso del processo elettorale. L'Assemblea del Senato si accorge ora di essersi mossa tardi e male nel rimediare a un *vulnus* costituzionale evidente fin dall'inizio della legislatura. Non era bastato il ricorso immediato del primo dei non eletti nella lista del Popolo della Libertà nella ripartizione Europa, che dimostrava e denunciava l'assenza di un requisito fondamentale nella candidatura della persona in questione: la residenza fissa all'estero. Non era bastata, nel giugno del 2008, la prima richiesta d'arresto avanzata dal giudice per le indagini preliminari di Roma, Luisanna Figliola, con la sconcertante rivelazione di tutta una trama a Bruxelles, volta a nascondere l'ineleggibilità del candidato ricorrendo a un molteplice falso in atto pubblico, in cui si profila anche una corresponsabilità di autorità diplomatiche e consolari, come le intercettazioni telefoniche ampiamente documentano. Non era bastata alla maggioranza della Giunta delle elezioni, che nel settembre 2008 votava contro l'esecuzione dell'ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari, la incredibile lista di imputazioni che andavano dall'attentato ai diritti politici dei cittadini e dalla falsificazione dei documenti di residenza al concorso in falsità ideologica e concorso in abuso d'ufficio. Non era bastata poi, l'anno scorso, finalmente la decisione unanime della Giunta delle elezioni che proponeva la destituzione del senatore e autorizzava l'esecuzione del mandato d'arresto. Non era bastato neppure tutto questo ad impedire che una maggioranza garantista ad oltranza in quest'Aula insensatamente ribaltasse la proposta della Giunta delle elezioni e votasse il cosiddetto ordine del giorno De Gregorio, per congelare la decadenza del senatore e le conseguenze pratiche del caso nella provvidenziale attesa di un rinvio a giudizio e magari di una sentenza passata in giudicato. in giudicato. È dovuto arrivare un secondo ordine d'arresto, corredato stavolta dell'imputazione di sordidi crimini di riciclaggio internazionale e associazione a delinquere, per un sussulto di coscienza e senso di responsabilità e urgenza. di responsabilità e urgenza. Più che opportuna era, pertanto, la mozione del gruppo del Partito Democratico, respinta ieri in quest'Aula con lo stesso puntiglioso spirito prevaricatore di sempre, che impegnava il Senato a revocare l'infausto ordine del giorno De Gregorio. In altre parole, per poche ore si è voluto sospendere la mozione di sospensione, invece di sospendere il già dimissionario senatore: un farraginoso guazzabuglio procedurale, regolamentare e interpretativo che fa a stracci la logica e la serietà del legislatore agli occhi dell'opinione pubblica nazionale, e purtroppo anche internazionale, come ha ricordato ieri la presidente Finocchiaro. La discussione di quella mozione sarebbe stata un passo utilissimo per fissare i contorni reali del caso, e per certi versi poteva costituire un'azione propedeutica ad affrontare un altro impegno, un'altra sfida, un'altra prova che ci attende e alla quale ben pochi stanno pensando: lo scrutinio delle credenziali atte ad avvalorare la piena legittimità del successore di Di Girolamo, il primo dei non eletti nella lista del Popolo della Libertà nella ripartizione Europa della circoscrizione Estero. Attenti ad evitare dubbi, incertezze e pressappochismo di valutazione, perché arriva già - come ha ricordato il presidente D'Alia - qualche poco rassicurante avvisaglia di possibile controversia e di possibile contenzioso in materia. Si tratta di passi prudenti e necessari per scongiurare che con il polverone della vicenda si gettino ombre immeritate sulla legittimità e onorabilità di tutti gli eletti all'estero: di infami calunnie, sempre smontate ma pur sempre dolorose, ne ho anche esperienza personale sulla mia pelle di eletto e rieletto all'estero; di scongiurare, ancora, che su un passaggio così triste per la nostra democrazia si innestino le speculazioni estremistiche, populiste, reazionarie, di quanti propongono l'abrogazione *tout court* dell'esercizio del diritto costituzionale di voto di voto dei cittadini italiani dovunque risiedano nel mondo.

hanno una rilevanza costituzionale e figurarsi se non ce l'hanno quanto all'andamento dei lavori dell'Aula del Senato della Repubblica. un'assemblea del Gruppo di maggioranza dell'Aula del Senato in parallelo con lo svolgimento della seduta dell'Aula e non credo che i colleghi delle opposizioni intendano prendere la parola,

La richiesta del presidente Rutelli è condivisa dal Gruppo dell'Italia dei Valori che, in mancanza di una sospensione della seduta, abbandonerà immediatamente l'Aula. Stiamo parlando di una cosa seria, per cui se i senatori di piano istituzionale rimanere qui. Stiamo parlando delle dimissioni di un parlamentare indagato per fatti gravissimi e tra l'altro appartenente al Gruppo di maggioranza.

gradiremmo la presenza del Governo in forma costante. Ora è fortunatamente rientrato il

la vicenda che riguarda il senatore Di Girolamo si sarebbe conclusa con un applauso dei senatori della maggioranza, a giubilare un comportamento che veniva ritenuto nobile e conclusivo di una vicenda che ha peraltro profili di delicatezza politica, istituzionale e costituzionale che i colleghi hanno già illustrato e che torneremo a illustrare nel tempo che ci separa dalla decisione. Non potevamo prevedere, neanche nelle nostre più pessimistiche ipotesi, che al giubilare della maggioranza (con un applauso vivo e prolungato, come sarà scritto nei resoconti), sarebbe seguito il fatto che che non uno dei colleghi del PdL - salvo la senatrice Barbara Contini - sarebbe rimasto in quest'Aula a seguire un dibattito che dovrebbe invece interessare, il Senato. In queste condizioni, per lo stesso decoro dei nostri lavori, mi associo alla richiesta dei colleghi per la sospensione dei lavori.

di chi prende atto delle dimissioni di un collega per un atto politico è totalmente inaccettabile e dimostra a quale livello il dibattito viene portato dalla sinistra.

(diversamente dall'opposizione). Capisco pure che in questo momento è evidente che la maggioranza non sono io, che rappresento un'assoluta minoranza in Aula, però, presidente Zanda, mi faccia mettere in fila almeno cinque parole. Se, invece, i colleghi insistono,

ai sensi dell'articolo 59 del nostro Regolamento, nonché ai sensi dell'articolo 64 della Costituzione. Il Governo ritiene di non essere presente per sua scelta: noi riteniamo che, avendo un Gruppo chiesto la presenza del Governo in Aula,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi è sicuramente un giorno increscioso per quest'Aula. Le dimissioni di un componente dell'Assemblea per motivi oggettivamente gravi

riflessione. La riflessione che intendo sviluppare serenamente con gli altri colleghi non riguarda

delle candidature e dei rischi di infiltrazione mafiosa nella selezione delle classi dirigenti del Paese, evocato

apre lo spazio per questa riflessione. La politica ha bisogno di atti concreti e non di operazioni di propaganda, proprio perché tutti siamo consapevoli della della pervasività delle organizzazioni criminali e del rischio di inquinamento nelle rappresentanze elette. Le mafie sono la morte della democrazia e della politica. allora la politica, per difendere il proprio ruolo nobile, deve riuscire a trovare dei momenti condivisi di risposta seria, coerente e concreta. Ho apprezzato

se pensiamo che poco tempo fa - saranno due o tre mesi - in un'altra Aula, nell'altro ramo del Parlamento, altro imputato di reati altrettanto gravi, se non più gravi, per il quale era stato chiesto l'arresto è stato invece protetto dal voto assembleare, per cui si è ritenuto di non accedere alla richiesta della magistratura (quella

rigettando la richiesta di arresto che riguardava il reato di concorso in associazione mafiosa e addirittura consentendo la permanenza nella compagine governativa di questo parlamentare. Queste due incoerenti posizioni pongono un problema.

per spirito di propaganda positiva (la mia non è una critica, capisco l'ansia di comunicare al Paese), è venuto e continua a dirci che, negli ultimi due anni, sono stati confiscati alla mafia beni per 7 miliardi di euro. È chiaro che si tratta di una comunicazione propagandistica: nella relazione al Parlamento sulla consistenza dei beni confiscati,

è pari ad un valore di 220 milioni di euro; altro che 7 miliardi di euro. Lo abbiamo però interpretato come un messaggio propagandistico. Abbiamo ritenuto che fosse un messaggio propagandistico quello del Governo quando di aver inasprito il regime del 41‑*bis*; sappiamo benissimo che l'inasprimento del 41-*bis* è un'iniziativa parlamentare frutto di un emendamento presentato da tutti i partiti presenti nel Parlamento, e non del Governo, che non aveva proposto questa misura. Abbiamo ascritto al bisogno di propaganda il fatto di sostenere che il Governo avrebbe inserito la norma sull'applicazione delle misure di prevenzione disgiunte dalla prevenzione personale, ossia nel senso di inseguirela pericolosità del bene; anche questa non è stata un'iniziativa del Governo, ma un'iniziativa parlamentare mutuata da un disegno di legge presentato dall'Italia dei Valori. Abbiamo purtroppo dovuto constatare - ecco i segnali contraddittori il fatto che non si sia ancora riusciti a far approvare dal Parlamento l'introduzione del reato di autoriciclaggio. Lei ricorderà, signor Presidente, che a gennaio del 2009, alla vigilia del voto, si operò un stralcio; da quel momento non si è riusciti a portare in Aula la proposta di introduzione del reato di autoriciclaggio, strumento necessario, ritenuto altamente significativo per il contrasto alla

(che risale al 1931) all'articolo 29, ossia l'interdizione a ricoprire cariche pubbliche (per condanne superiori a cinque anni si prevede l'interdizione perpetua, mentre per condanne da tre a cinque anni l'interdizione temporanea sino a cinque anni). Ciò che viene presentato come un'innovazione è un arretramento rispetto a quello che già esiste. Oggi c'è un fatto nuovo che io, signor Presidente, vorrei richiamare all'attenzione Lo scorso 18 febbraio la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle mafie ha approvato un codice di autoregolamentazione,

è possibile che la politica non si renda conto che non può opporre il silenzio a ciò che la Commissione antimafia all'unanimità ha proposto alla politica, che non si renda conto che deve dare una risposta concreta a una sollecitazione che riguarda i rischi di infiltrazioni mafiose nelle candidature per la selezione delle classi dirigenti? I partiti dovrebbero manifestare concretamente adesione. Ovviamente, noi come Commissione antimafia non possiamo imporre: offriamo ai partiti l'opportunità di sottoscrivere e aderire al codice di autoregolamentazione. Ma è mai possibile che le forze politiche ostentino un fragoroso silenzio su questa proposta? Noi, come Italia dei Valori, vi abbiamo dato seguito seguito inserendo quel codice di autoregolamentazione nello statuto e comunicando l'elenco dei nostri candidati alla Commissione antimafia. La politica deve dare al Paese un segnale, un segnale forte e condiviso che ci veda tutti uniti, come lo siamo stati in Commissione antimafia. Si pronunzi

di livello di contrasto, che ci veda uniti nella condivisione di alcuni principi. Salviamo la politica, perché salvando la politica salviamo la democrazia. Cogliamo l'occasione di questo dibattito in un giorno increscioso e facciamone un momento positivo di assunzione di responsabilità. Che si alzi da questa Camera alta del Parlamento un comune segnale al Paese: siamo uniti contro le mafie, vigileremo sulle candidature, non candideremo coloro che sono imputati di fatti di mafia, così come prevede il nostro codice di regolamentazione. Si abbia il coraggio di fare questo. È questo che vuole il Paese, è questo che noi dobbiamo al Paese, nell'interesse del Paese.

perché questo dibattito è rilevante per il Senato e per i suoi componenti. Credo che noi oggi dobbiamo, signor Presidente, fare ammenda come istituzione della vicenda precedente, ovverosia di quell'artificio che ingloriosamente fu adottato quando ci siamo occupati precedentemente dell'eleggibilità del senatore Di Girolamo. Credo sia stata un'espressione di partigianeria, signor Presidente. Credo che si sia trattato di una pagina non positiva per il Senato e penso che l'occasione odierna, anche se non ha preso il binario giusto dal punto di vista formale, può portarci nuovamente sul binario giusto.

a sua volta l'autorità del Senato. Vede, signor Presidente, il vento in politica cambia frequentemente le circostanze nelle quali delle maggioranze politiche si reputano forti o addirittura blindate possono mutare. Non mi auguro che nel nostro Paese ritornino le condizioni che abbiamo conosciuto in altre stagioni politiche e, proprio per questo, mi auguro che sappiamo distinguere nelle decisioni istituzionali, fatta la tara della passione politica dello schieramento, la partigianeria politica dalle esigenze delle istituzioni. In questo caso, penso che quando il Senato si trovò di fronte - mi si passi l'espressione - alla falsa alternativa se arrestare un collega

- ma avevamo votato a favore della decadenza, perché erano evidenti già allora le condizioni della ineleggibilità del collega Di Girolamo. oggi ci troviamo in una condizione che ci suggerisce di ritornare su quella fase della vita parlamentare, non solo per lasciarlo agli atti del Parlamento e nei verbali della nostra Assemblea. Il senatore Augello, ora passato ad un incarico di Governo, in un'intervista rilasciata pochi giorni fa ha ricordato quella vicenda e il suo dissenso;

a quello che lui definisce "un conflitto notevole con il mio Capogruppo, quel giorno e in quelli precedenti", richiamando per parte sua - il senatore Augello - la coerenza della posizione che aveva assunto con il senatore Follini in seno alla Giunta competente, che non si è sentito, assieme ad alcuni altri colleghi, di sconfessare poi in un voto d'Aula che, per l'appunto, Presidente, rispondeva ad una istanza partigiana, ad una decisione politica: una maggioranza che si sente forte blinda un suo esponente, non se la sente di prendere atto del fatto che un'istanza giuridico-regolamentare è invece fondata e conviene, anziché fare una battaglia pro o contro l'arresto di un collega senatore, fare una battaglia per constatare invece le condizioni della sua ineleggibilità. Signor Presidente, questa riflessione oggi non voglio farla con riferimento alla vicenda giudiziaria. Dobbiamo recare rispetto all'azione della magistratura e anche alla decisione del collega Di Girolamo che a tale procedimento si è affidato, si è rimesso, rinunciando al proprio mandato parlamentare.

su questa materia, ma sulle prerogative del Senato e anche sulla vicenda della legge per l'elezione dei rappresentanti degli italiani all'estero. Lo hanno fatto alcuni colleghi e altri credo che lo faranno, e non è questa soltanto la circostanza in cui lo potremo fare, però carissimi colleghi, signor Presidente, è evidente che quella legge non solo zoppica, ma ha dimostrato tutte le sue falle. Infatti, in realtà il Parlamento e le diverse maggioranze parlamentari, tutti noi, ci siamo presi la responsabilità di varare una normativa sul diritto di voto degli italiani all'estero corrispondente ad una aspettativa, in particolare propugnata molto onorevolmente dal collega Tremaglia, che era fondata su un dibattito iniziato cinquant'anni fa. La natura e l'organizzazione del voto degli italiani all'estero riflettono un'impostazione vecchia, iniziata cinquant'anni fa, che rispondeva ad un'esigenza giusta, che è stata declinata - come dicevo - in modo fallace dal punto di vista normativo ed organizzativo, ma fondamentalmente vecchia nell'interpretazione della natura e degli interessi delle nostre comunità all'estero: il che è stato anche dimostrato in parte dall'esito di alcuni passaggi elettorali.

non l'ironia di cui spesso sono destinatari per il fatto che sono pendolari in circoscrizioni impossibili: pensiamo alla circoscrizione che unisce l'Africa, il Medio Oriente, l'Antartide, l'Asia e l'Oceania

Il problema che si pone è propriamente quello democratico, per una grande Nazione, signor Presidente, di circa 60 milioni di abitanti, che ha molte decine di milioni di connazionali nel mondo: ne siamo profondamente orgogliosi, li vogliamo far partecipare alla vita della nostra Nazione, alle elezioni democratiche che deeterminano la formazione del Parlamento della Repubblica. Ma non ci possiamo più nascondere la realtà: il diritto di voto può andare, Presidente, a nostri connazionali che non parlano la lingua italiana? Quanti sono gli elettori riconosciuti che non possono partecipare democraticamente alla formazione del consenso perché non parlano la lingua italiana? Vogliamo affrontare questo argomento? Prescindiamo, però, dal tema di fondo, colleghi, che è alla base della democrazia, ossia *no taxation without representation*. Si può non pagare le tasse e votare? È un tema, ovviamente, che ha bisogno di una soluzione generale. La mia conclusione, Presidente, riguarda due punti. Per il malcostume politico è legato al fatto che alcune persone si candidano non avendo le prerogative stabilite dalla legge. Presidente, mi permetto di fare

siete sicuri che alcune scelte che si fanno dal punto di vista etico, politico e istituzionale in quest'Aula rimarranno intatte?

dell'istituzione con la politica, ma anche dell'istituzione con l'opinione pubblica e con i fondamenti di una lealtà verso le istituzioni di cui tutti noi, pur nelle difficoltà che conosciamo, dobbiamo essere portatori. a lei con grande rispetto e grande fiducia: il Parlamento ha bisogno, in entrambi i lati di quest'Aula, di dismettere non la passione politica e la divisione sui grandi temi che ci contrappongono in politica, bensì la partigianeria. La pagina che abbiamo conosciuto con la precedente falsa alternativa posta tra decadenza o arresto del collega Di Girolamo

Penso che da questa vicenda si possa uscire positivamente solo se il Senato fa marcia indietro rispetto a quella pagina. Riconosciamo al senatore Di Girolamo la dignità del suo gesto di oggi; affidiamo alla magistratura il compito di accertare le gravissime circostanze su cui l'inchiesta si sta sviluppando, ma salviamo il Senato della Repubblica nella sua capacità di discernere, signor Presidente, tra un momento in cui la maggioranza si blinda ciecamente e un momento in cui, invece a decidere - e spero che da oggi ci muoveremo in questa direzione - sarà sempre e solo l'interesse dell'istituzione, anche se scomodo, per la nostra parte o per un'altra, a un'altra, a tutela dell'istituzione. Lei è garante di questo ed io le rinnovo la fiducia perché in questa direzione lei guidi il Senato della Repubblica. *(Applausi

ma non c'è nemmeno un Governo che assuma l'iniziativa per la cacciata dei nemici della Repubblica in maniera seria, molto più seria di quella che abbiamo sentito annunciare dalle liste per le

preferirei sottrarmi alla loro vista piuttosto che essere oggetto di sguardi di disapprovazione». Oggi noi dovremmo poter dire, o meglio il senatore Di Girolamo aveva l'occasione di dire: «Se mi accorgessi di essere, anche a torto, gravemente sospettato e disprezzato dai miei colleghi senatori italiani, preferirei cercare, pretendere, trovare ogni possibilità di difesa e di discolpa davanti a loro, piuttosto che essere oggetto di sguardi di compatimento e di abbracci di umana solidarietà

presentarsi ieri alla Giunta delle immunità per tutelare non solo il suo di onore, ma anche il nostro, del Senato, a riferire, nell'ambito del procedimento sulla sua richiesta di arresto, soprattutto in merito agli aspetti di rilevanza politica; quelli che oggi ci interessano. E' di ieri l'allarme della Commissione antimafia. Il senatore Di Girolamo avrebbe potuto chiarire il rapporto tra la sua dichiarazione patrimoniale depositata qui in Senato e l'ingente disponibilità di beni e mezzi finanziari che emerge dai dati di indagine consegnati a questa istituzione parlamentare. E avrebbe potuto - e dovuto, a mio avviso discolparsi, respingere e fornire elementi contro l'accusa a mio giudizio più grave: quella di broglio elettorale coordinato e organizzato dalla 'ndrangheta. Ritengo che il broglio sia tra le peggiori offese alla democrazia.

onorando l'articolo 66 della Costituzione) ci dice che esistono delle regole da cambiare. Sì, ci sono delle regole da cambiare. Essere all'altezza della Costituzione è sempre difficile, però in questi anni è stato difficilissimo rintracciare una decente applicazione dell'articolo 66 della Costituzione. Dobbiamo cambiare i tempi delle nostre decisioni. Ci sono oggi casi che pendono davanti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari a quasi due anni dall'inizio della legislatura.

in un contesto che risentiva ancora fortemente degli abusi subiti dal Parlamento in epoca fascista e che, dunque, deponeva per una incondizionata affermazione del principio di autodichia (cioè di giustizia su noi stessi, quella che è prevalsa nell'articolo 66 nell'articolo 66 della Costituzione) - capiva che il problema di garantire l'effettiva tutela delle minoranze contro il pericolo di un giudizio condotto solo con criteri politici doveva ritenersi "non solo eventuale, ma concreto, e che esso tende a divenire sempre più grave via via che la lotta politica assume carattere di maggiore asprezza". Torniamo a quella riflessione, soprattutto in relazione alla composizione su base maggioritaria di questo Parlamento. Offriamo un'istanza di appello a una nostra a una nostra più rapida decisione. Oggi la Corte costituzionale può essere sicuramente questa importante, lineare e trasparente istanza di appello. Nella imperfetta giustizia degli uomini sarà una giustizia più informata a un'idea moderna di democrazia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, questa è una giornata che è e rimarrà, purtroppo, sotto il segno di un avvilente imbarazzo: imbarazzo per la storia, la vicenda e imbarazzo per la dignità stessa del Senato. Voglio ricordare le espressioni che all'inizio il GIP aveva usato per chiedere l'autorizzazione all'esecuzione degli arresti domiciliari: «In spregio alle istituzioni e senza alcun rispetto per il corpo elettorale e per i diritti politici del cittadino, con una serie incredibile di inganni ha impedito di fatto che gli elettori potessero manifestare le proprie scelte essendo stati indotti in errore». Ma, al confronto con queste espressioni, quello che siamo venuti a sapere dopo è molto peggio. È vero che si tratta di cose che non sono state ancora accertate dall'autorità giudiziaria, però sapere aiuta, in quanto ci permette di esprimere un giudizio, e ciò che sappiamo oggi è assai più grave di quello che era contenuto nelle accuse del GIP. È emersa un'ombra oscura sul voto all'estero. Ha ragione il senatore Micheloni a ricordare che ci sono tanti parlamentari che sono stati eletti in maniera giusta e corrispondente alla volontà dei cittadini, ma resta un'ombra di dubbio. Ha ragione, sempre il senatore Micheloni, a ricordare che le radici di questo malaffare non sono all'estero, ma sono in Italia, radicate nel tessuto del rapporto tra affari, politica e anche criminalità organizzata. È stato imbarazzante il rifiuto dell'Aula nei confronti delle conclusioni della Giunta delle elezioni che aveva condotto una sua indagine, aveva ascoltato i testimoni, aveva vagliato delle notizie aveva espresso una proposta favorevole alla decadenza del senatore sospettato in questo caso. L'Aula ha voluto rifiutare quelle deduzioni questo è veramente un motivo di riflessione per l'intera Assemblea. Imbarazza, infine, l'atteggiamento minimizzatore del dimissionario, il quale si presenta il capo cosparso di cenere, ma in realtà tenta di ridurre al minimo e alle minori le accuse che gli vengono mosse. Si difende sulla questione delle fotografie, ma non dice una parola ‑ e questo è un segno di imbarazzo per lui stesso ‑ sulle terribili espressioni che usano le persone che parlano con lui e che abbiamo letto, riferisco ad un individuo che vive ai margini della legge, che si permette di dire ad un senatore: «Tu sei una cosa mia. Faccio di te quello che voglio».

che se ne va: non bisogna infierire, però bisogna mantenere saldo il ragionamento. Non possiamo accettare l'ipocrisia di prendere per buone le dimissioni senza pronunciarci sulla decadenza, della quale la Giunta stessa, all'inizio, aveva parlato: accettare le dimissioni è una sorta di uscita di servizio malaccorta, scivolosa, che esprime il disagio, ma lo nasconde. Per uscire dall'imbarazzo, onorevoli colleghi, è fondamentale

alla dignità democratica, ed è proprio in questo senso che il Gruppo dell'Italia dei Valori si muoverà. Presidente, questa storia per me sta dentro la cronaca, che a sua volta sta dentro le date,

la proposta di accoglimento del ricorso in merito all'elezione del senatore Di Girolamo.

Vorrei ricordare a me stesso quale poderosa accelerazione avremmo determinato se fossimo rimasti fermi al pronunciamento della Giunta di oltre un anno fa, risparmiando al Senato le le vicende di cui questi giorni sono piene le cronache, e rispettando una conclusione a cui le diverse parti politiche avevano collaborato

a dispetto del cambiamento di umore, di clima dell'Aula, determinato quel giorno sotto la sua Presidenza. Voglio ricordare che nell'opinione pubblica questa vicenda allude alla zona grigia che corre tra le istituzioni e la criminalità, evocando quindi problemi di straordinaria delicatezza e intensità politica. Ovviamente, sarà la magistratura a chiarire, ma noi non possiamo sfuggire ai problemi politici che ci vengono posti, ed io ne vedo due in particolare. Un problema riguarda il senatore Di Girolamo e i suoi conti con la giustizia: problema che Di Girolamo ha affrontato con un gesto che merita da parte mia rispetto, e non lo dico in modo rituale. L'altro problema riguarda noi: liquidare la presenza del senatore Di Girolamo in questi mesi e il voto con cui l'Aula gli ha consentito di rimanere per un anno e più, come fosse un fatto minore, una circostanza piccola e occasionale, credo sia sbagliato da parte di tutti, ma è tanto più inaccettabile da parte di chi ha accompagnato e sostenuto il suo percorso politico. Non stiamo parlando di un figlio di N.N.; stiamo parlando di un senatore che è stato parte di un procedimento politico che il dibattito di questa mattina ha largamente richiamato. La Giunta in tutti questi mesi è stata vincolata - come veniva ricordato prima - da un ordine del giorno che cammin facendo si è rivelato per quello che era ed è: senatore Rutelli ha benevolmente parlato di un atto di partigianeria politica; io penso che sia stato piuttosto un gioco delle tre carte, e come tale si rivela. Ora occorre guardare oltre questa vicenda e cercare, per quanto è possibile, di correggerne gli effetti. Voterò ovviamente per accogliere le dimissioni del senatore Di Girolamo, ma segnalo che da questa storia, da questa brutta storia, signor Presidente, possiamo uscire con dignità, decoro e potremmo uscirne anche con limpidezza se fossimo capaci di guardare dentro lo specchio degli errori che complessivamente abbiamo fatto. Ma per questo occorre rimettere le coscienze e le istituzioni lungo la stessa linea. La maggioranza ha scelto oggi di archiviare Di Girolamo e di assolvere se stessa; noi, all'opposto, votiamo per le sue dimissioni perché resti ferma da parte nostra la condanna dell'arroccamento e dello spirito di parte, che ha portato il Senato fin qui. Queste sono le ragioni del voto con il quale accogliamo le dimissioni del senatore Di Girolamo.

e delle immunità parlamentari, mi sono permesso di dire che abbiamo allestito il patibolo mediatico e che era pronta la ghigliottina per il senatore Di Girolamo. Stamattina eseguiremo la condanna e il senatore Di Girolamo diventerà il signor Nicola Paolo Di Girolamo, verrà arrestato e risponderà alla giustizia dei reati che gli vengono contestati. Ma, cari colleghi, sono d'accordo con il senatore Pardi, sul fatto che questa sia una pagina non fulgida delle istituzioni parlamentari. sono d'accordo, non tanto e non solo per ciò che è Nicola Paolo Di Girolamo (e, peraltro, ancora mi chiedo chi è questo signore, visto che il GIP di Roma, che ci ha chiesto il suo arresto, prima lo definisce il capo e il promotore di un'associazione a delinquere di stampo transnazionale finalizzata a commettere un'infinità di reati gravissimi e poi conclude dicendo: «Il Di Girolamo costituisce solo uno strumento per consentire al gruppo criminale di fare ingresso nella porta principale delle istituzioni dello Stato»; «Che di Girolamo non conti nulla o meglio che debba essere un mero *nuntius* delle scelte operate dal gruppo, in primo luogo di Mokbel, emerge chiaramente»). Già questo mi fa pensare che il GIP, che ha perfettamente ragione e al quale faremo un monumento, è un po' confuso: Nicola Paolo Di Girolamo? Un criminale davvero, cioè il capo, il promotore di questa organizzazione criminale, o una persona che ieri mi sono permesso di definire con un'espressione milanese, che non userò in quest'Aula, perché non mi va di ripeterla, ma diciamo che conta poco o nulla, e che probabilmente non è il capo dell'organizzazione criminale? Mi sono permesso di ricordare ieri anche i tempi dell'ordinanza del GIP. Il pubblico ministero presenta le sue 1.600 pagine di indagine al GIP il 13 agosto 2009 e dice al GIP che nel Senato c'è una persona pericolosa, una persona che si è fatta eleggere con i voti della 'ndrangheta, il braccio operativo istituzionale della 'ndrangheta. Il GIP firma l'ordinanza il 3 febbraio del 2010 e ce la notifica il 22 o il 23 febbraio 2010: aspetta sei mesi per emettere un'ordinanza su un criminale che passava in queste Aule e viveva nelle nostre Commissioni. Se fosse - e noi siamo sicuri che lo è - un criminale, credo che il GIP avrebbe dovuto accelerare al massimo questa contestazione e fornirci quegli elementi probatori che un anno fa non ci fornì, perché quando decidemmo un anno fa, tutti assieme, con votazione unanime, unanime, il rigetto degli arresti domiciliari di Di Girolamo - votazione unanime su proposta conforme della Giunta - gli unici elementi probatori a carico di Di Girolamo erano una serie di «frasettine». Poi scopriamo, oggi,

di quegli elementi probatori ci fu fornito nel 2008 e nella richiesta del GIP del 2008 non si accenna minimamente ad elementi probatori che scopriamo ora. Allora mi chiedo: perché il GIP non ci ha fornito un anno fa quello che inizia a fornirci oggi?

Sono solo riflessioni, perché la ghigliottina è già allestita e abbiamo già il patibolo pronto e bello caldo! e bello caldo! Colleghi, credo che sia una pagina amara: amara per i discorsi un po' paludosi che ho sentito, dove si cerca di scaricare la responsabilità di qua o di là, quando la responsabilità è anche di una magistratura che di fronte ad un procedimento per falso in certificato MAZZATORTA *(LNP)*. L'ordine del giorno De Gregorio diceva di sospendere in attesa che la magistratura facesse il suo corso su un procedimento di falso per un certificato anagrafico: parlamentari, lo scorso anno, in tre giorni ha sentito tutti i testimoni della vicenda e in tre giorni si è pronunciata. Se il tribunale di Roma si fosse pronunciato in primo grado su Di Girolamo sul reato di falsità in certificato non dico in tre giorni, ma in tre mesi,

Allora forse - forse, ma sicuramente non sarete d'accordo - una parte di responsabilità va anche ad una magistratura ad orologeria. Ecco perché, alla fine di questa vicenda poco edificante, che dimostra che forse ci siamo piegati più alla strumentalizzazione mediatica che ad una verifica concreta delle situazioni, anche noi voteremo a favore dell'accettazione delle dimissioni, ghigliottineremo Di Girolamo e andremo avanti.

è mancato - e mi permetto di proporlo io - è la contestualizzazione della vicenda Di Girolamo e del suo esame parlamentare. Questa, infatti, non può essere scissa da quello che è stato l'andamento dei nostri lavori e anche dagli atteggiamenti politici e istituzionali della maggioranza e del Governo in questi due anni. in questi due anni. Lo abbiamo detto molte volte da questi banchi e adesso il fatto di dirlo sinteticamente probabilmente farà sembrare più *tranchant* la mia descrizione: abbiamo assistito in questi anni ad una demolizione sistematica delle attribuzioni, del ruolo, della funzione e della stessa dignità del Parlamento, innanzitutto come luogo centrale di un sistema costituzionale che vede appunto una democrazia parlamentare instaurata nel nostro Paese. Probabilmente la demolizione avvenuta in maniera più sotterranea, ma non per questo meno grave sotto il profilo degli effetti prodotti, è stata la riforma elettorale: nel momento in cui il Parlamento non viene composto da soggetti che rispondano agli elettori e che dagli elettori sono eletti, bensì da persone che vengono nominate dai segretari di partito, in quel momento il Parlamento perde la propria funzione e anche la propria capacità di essere non soltanto potere indipendente e autonomo in un sistema di poteri indipendenti e autonomi legati da un sistema di *checks and balances*,

La seconda demolizione si è abbattuta sulla funzione parlamentare. Come abbiamo sottolineato tante volte, l'abuso dei decreti-legge, dei maxiemendamenti, dei voti di fiducia e delle ordinanze della Protezione civile

L'ordine del giorno De Gregorio è la *species* con la quale si è incarnata la volontà di abbattere questa prerogativa e questa assoluta sovranità del Parlamento. Non c'entra niente l'accanimento nei confronti del senatore Di Girolamo, nei riguardi del quale non ho alcun motivo di astio e neanche di antipatia. In questo caso, con l'ordine del giorno De Gregorio si spossessa il Parlamento di un'attribuzione esclusiva, peraltro molto diligentemente elezioni e delle immunità parlamentari, e si stabilisce che la permanenza del senatore Di Girolamo, oggi, e dei molti altri che verranno nella storia repubblicana è appesa alla decisione dei giudici ordinari. ultimi - nell'ambito di un giudizio che nulla ha a che vedere con quello sull'ammissibilità e sulla verifica dei presupposti, ma ha tut'altre caratteristiche, tutt'altro oggetto, tutt'altre regole e tutt'altre attribuzioni e competenze - decideranno se oggi il senatore Di Girolamo e, domani, i mille deputati e senatori che si troveranno in condizioni analoghe potranno o non potranno sedere in Parlamento.

che viene definito ai livelli più alti - e, in particolare, dal Presidente del Consiglio - nel quale si contesta sempre l'agire della magistratura, anche quando decide sull'ammissibilità di una lista elettorale; poi, però, si consente alla magistratura di determinare la composizione delle Camere.

con la totale indifferenza per ogni valore, principio e regola. Di qualunque genere. (*Applausi dal Gruppo PD*). Si decide sempre, comunque e soltanto rispetto a ciò che in quel momento torna più utile! La coerenza non è mai un metro dell'agire politico e istituzionale:

la cifra che muove e determina gli atteggiamenti. A mio avviso, questo non è il ruolo e l'essenza della politica né quello delle sue classi dirigenti. Al contrario, la politica dovrebbe avere l'ambizione - visto che ne ha il privilegio - di guidare il Paese, e non di assecondarlo piegandosi e modellandosi anche nelle pieghe meno onorevoli - lasciatemelo dire - dei sentimenti che pure nel popolo esistono e possono albergare, e che anzi vengono assecondati. Una volta vi dissi da questi banchi che rimproveravo al presidente Berlusconi di aver fatto ammalare l'anima dell'Italia: lo ribadisco, ed è la conseguenza di questo modo di procedere, che fa gravi danni e, lasciatemelo dire, fa anche molto modesti i vostri risultati.

politica, sostenuta da un supremo disprezzo per le forme, i valori, gli strumenti, le regole repubblicane. Oggi in quest'Aula tutto ciò assume la *species* dell'ordine del giorno De Gregorio. Voglio dire una cosa con estrema chiarezza, signor Presidente, perché affido a lei e alle sue decisioni l'autorevolezza e la dignità di quest'Aula. Noi ora voteremo le dimissioni del senatore Di Girolamo, e voteremo a favore, ma dopo voteremo la revoca dell'ordine del giorno De Gregorio *(Applausi dal Gruppo PD)*, perché questa è l'unica possibilità che abbiamo per restituire a quest'Aula la dignità e l'autorevolezza che in questi giorni, e ancora stamattina con quell'assenza, abbiamo visto da voi comprimere nell'Aula del Senato.

Presidente, colleghi, questa bruttissima pagina della storia del Senato poteva esserci evitata un anno fa dallo stesso senatore Di Girolamo e dalla maggioranza. Un anno fa erano emersi elementi tali che dovevano consentire di accedere alla richiesta giudiziaria, ovvero alle dimissioni del senatore Di Girolamo. Vede, signor Presidente, è sempre un problema di regole. È un problema di regole, perché quando esistono, siano esse formali o sostanziali, vanno rispettate sempre.

perché ha consentito di aggirare un voto precedente e soprattutto un parere che la Giunta delle elezioni aveva espresso. Ecco perché l'Italia dei Valori ritiene importante collegare le due cose. Ricordo che su quell'ordine del giorno si sono espressi l'anno passato i senatori Compagna, Orsi, Malan, Pastore, Vetrella, De Gregorio e Cuffaro: li inviterei a chiedere scusa all'Aula, perché l'hanno sottomessa ad un ordine del giorno veramente infame. Voteremo certamente per l'accoglimento delle dimissioni del senatore Di Girolamo, però ci associamo alla richiesta che ha avanzato il Partito Democratico: chiediamo di votare per la revoca di quell'ordine del giorno, che oggi non avrebbe neppure una ragione strumentale per rimanere in piedi.

Signor Presidente, in primo luogo voglio riprendere alcune considerazioni che ho già avuto modo di svolgere ieri in riferimento ai precedenti

quella scelta - la priorità delle dimissioni presentate dal senatore di Girolamo rispetto alle altre procedure in atto. Ho citato ieri, e riferisco ancora oggi, i precedenti,

e della decadenza dell'onorevole Crippa, di fronte alla sua decisione di dimettersi, con parole chiare e rigorose, anche per criteri di economicità delle procedure, mise in votazione le dimissioni del parlamentare che, peraltro, erano intervenute nel corso del dibattito e non in precedenza, come in questo caso. il presidente Napolitano motivò e illustrò la sua scelta alla Camera dei deputati. Analogamente si regolò il Senato sul caso del senatore Magri. L'allora presidente Pera, qui presente, in maniera analoga dette precedenza alle dimissioni rispetto alle discussioni che pure all'epoca si facevano. Così come accadde anche nel 2007 nel caso dell'onorevole Previti con dimissioni, mi pare, addirittura annunciate con una lettura da un altro collega in Aula, che il presidente Bertinotti,

la non condivisione di una drammatica scelta assunta e motivata oggi da Di Girolamo. Quindi, le dimissioni si collegano a questi fatti nuovi ben più gravi. Quando discutemmo parlavamo di indirizzi e quant'altro e anche alcune guarentigie furono da noi valutate, non dicendo no, ma sospendendo quella decisione perché una contestazione di indirizzi avrebbe potuto determinare un arresto che ci apparve in quel momento, di fronte a quelle (non alle contestazioni di oggi), una conseguenza eccessiva. Ieri non ho ascoltato l'intervento svolto da un collega in quest'Aula che so essere stato particolarmente insultante. Ebbene, ho riletto il mio intervento di ieri

del Partito Democratico, eletto in Australia, fa riferimento ad un'inchiesta giornalistica che riguarda le modalità di elezione, le contestazioni, i plichi. So di essere stato insultato e ribadisco al senatore Randazzo che non l'ho offeso, che non sono giunto a conclusioni e che è in corso, come lui stesso pare abbia detto, un'inchiesta giudiziaria. Attenzione, allora, ad invocare il rispetto delle regole perché non so se tutti da quella parte dell'Aula sono in grado di invocare il rispetto delle regole.

Non ho tratto conclusioni ieri, non ne traggo oggi. Mi rammarico degli insulti che lei, senatore Randazzo, ha proferito e che respingo al mittente invitandola ad accettare ed attendere serenamente il giudizio sui possibili brogli che in Australia si sarebbero verificati.

non voglio ricordare solo le elezioni politiche: potrei ricordarle le elezioni del Friuli-Venezia Giulia, le elezioni della Sardegna, le elezioni di Roma, le elezioni dell'Abruzzo, le elezioni amministrative dello scorso anno, i cui risultati hanno dato e danno la maggioranza al centrodestra in questo Paese, non certo a voi, nemmeno dove

lunedì «la Repubblica», nell'ennesimo sondaggio, dava dieci punti di vantaggio al centrodestra. Poi, se qualcuno fa abusi sulle liste (perché questo è forse l'ultimo trucco: impedire di presentare liste per sferrare un colpo contro la democrazia) di questo discuteremo

(sicuramente qualche altro collega oggi qui in Senato, o perché membro del Governo o perché senatore, lo ricorderà), lei era deputata di una maggioranza che negli anni

non siamo certo qui a farci impartire lezioni da chi non ne ha titolo, visti i fatti dell'Australia, del collegio di Terlizzi che Vendola non aveva conquistato e tante altre questioni. Noi abbiamo deciso di votare a favore delle dimissioni di Di Girolamo e non stiamo qui a fare l'apologia di nessuno. Sarà la magistratura a fare quegli accertamenti. del rispetto, di cui ha parlato il senatore Rutelli e qualche altro collega: certo, rispetto è la parola che usiamo per una persona che oggi, dimettendosi, si chiude dietro le spalle le porte del Senato sapendo che oggi stesso si apriranno per lei le porte del carcere. È un percorso durissimo e doloroso. Ebbene, dietro questa scelta, che noi, con il nostro voto a favore delle dimissioni, sappiamo di determinare, c'è l'accettazione di un'inchiesta in corso e di accuse molto pesanti, che solo nei giorni scorsi il Senato ha conosciuto, che la Giunta competente ha appena istruito e cominciato ad affrontare e che le dimissioni di Di Girolamo consentono di discutere con decisioni ancora più appropriate. Concludo, cari colleghi, dicendo cosa potrà dire il Paese fuori di qui: capirà che c'è qualcuno che fa cavilli sulla sospensione della sospensione della sospensione; che c'è una persona che si dimette, che va in carcere, e noi votiamo a favore delle sue dimissioni. Questa è la verità che emergerà da questo dibattito. *(Applausi dal Fate anche cavilli: noi votiamo per le dimissioni sapendo cosa vuol dire e ce ne assumiamo la responsabilità. Non abbiamo nulla di cui rammaricarci e ci assumiamo davanti al Paese la nostra responsabilità. Votate anche voi per le dimissioni del senatore Di Girolamo!

Colleghi, vi prego di prendere posto perché dobbiamo passare alla votazione.

I senatori favorevoli ad accogliere le dimissioni premeranno il tasto verde al centro della postazione di voto; i senatori contrari premeranno il tasto rosso a destra; i senatori che intendono astenersi premeranno il tasto bianco a sinistra. Poiché si tratta di una votazione a scrutinio segreto, qualunque sia la scelta di voto effettuata, la luce che si accenderà sarà di colore neutro. Dichiaro aperta la votazione.

mozione del senatore D'Alia e delle altre che chiedevano la revoca del precedente provvedimento. Ringrazio i colleghi per aver richiamato la mia autorevolezza o un'eventuale mia iniziativa, ma non è un potere della Presidenza.

l'Aula si è pronunciata negativamente, bocciando tale richiesta. Quindi, l'Aula su questo argomento si è già pronunziata negativamente. C'è un voto, senatore D'Alia, mi dispiace: la richiesta è stata messa ai voti ed è stata bocciata. L'Aula è sovrana e su quella richiesta si è già pronunziata ieri in occasione della

la sollecitazione che è stata formalizzata anche questa mattina dalla presidente Finocchiaro, dal presidente D'Alia, fatta propria dal presidente Belisario. Voglio riepilogare l'andamento di questa vicenda che ha assunto i caratteri della complessità sotto il profilo procedimentale. Lei ieri, nel leggere l'esito della Conferenza dei Capigruppo, ha comunicato che si sarebbe passati all'esame delle mozioni qualora le dimissioni non fossero state accolte. Il voto sul calendario, a cui lei si riferiva poco fa, signor Presidente, riguardava la modifica dell'ordine cronologico e logico delle votazioni: sia la presidente Finocchiaro, sia il presidente D'Alia avevano motivatamente argomentato nel senso di ritenere che fosse necessario votare prima la revoca dell'ordine del giorno a suo tempo approvato, a prima firma De Gregorio, e dopo le dimissioni. Dopodiché le cose sono andate come sono andate. Noi riproponiamo questo tema e vorrei esporre, signor Presidente, le ragioni per le quali, a nostro modo di vedere, questa sua decisione la decisione che ha assunto la Conferenza dei Capigruppo a maggioranza è contrastante con il nostro Regolamento, in particolare con gli articoli 157 e 158. Questi articoli prevedono che le mozioni, una volta iscritte all'ordine del giorno, così come sono state iscritte seppur condizionatamente all'ordine del giorno, non sono più nella nella disponibilità della Presidenza, ma sono nella disponibilità dei proponenti e dell'Aula nel suo complesso, a meno che - è questo il punto, signor Presidente - le mozioni stesse non debbano intendersi precluse da una decisione precedente. - è questo il cuore dell'argomentazione che lei ha voluto ribadire poco fa - si può ritenere che, all'esito dell'accettazione delle dimissioni, quelle mozioni debbano intendersi precluse?

Quindi, esiste incompatibilità, signor Presidente, tra l'accettazione delle dimissioni e una votazione che accerti oggi nel senatore Di Girolamo del titolo giuridico per essere eletto senatore. Non vi è incompatibilità perché gli effetti che noi intendiamo rimuovere con la votazione delle mozioni sono ulteriori rispetto alle dimissioni. Non sono la stessa cosa. In sostanza, la parte che accomuna le due decisioni è che il senatore Di Girolamo non è più senatore da questo momento in poi, e questo è acclarato. Non è acclarato però quanto è accaduto o doveva accadere dalla data delle elezioni del senatore Di Girolamo fino ad oggi. Questo è il punto, signor Presidente. Lei non può impedire all'Aula del Senato di esprimersi a tale riguardo; ma

si produrrebbero due ulteriori effetti sostanziali. Il primo effetto si ricollega all'articolo 135-*ter* del nostro Regolamento.

di un anno fa, quella originaria, si intenderebbe automaticamente accolta. Il contenuto del comma 2 dell'articolo 135-*ter* del nostro Regolamento prevede appunto che la decisione della Giunta si intende accolta qualora 20 senatori non presentino una mozione di segno contrario. quindi, un effetto sostanziale ulteriore dall'accoglimento delle mozioni, e questa è una ulteriore ragione per la quale quelle mozioni devono essere votate. si produrrebbe un ulteriore effetto sull'attività successiva che saremo chiamati a svolgere fra poco in Giunta per determinare il subentro.

Magri. L'accertamento dell'assenza del titolo giuridico per l'elezione a senatore non è destinato a produrre necessariamente il risultato del subentro del secondo in graduatoria: potrebbe produrre, in teoria,

sulla base dell'attuale legge elettorale, ma era sulla base della vecchia legge elettorale, per esempio con l'attribuzione dei seggi con la quota proporzionale del sistema cosiddetto *mattarellum.*

che le ho detto. Una decisione che, peraltro, è stata autorevolmente sollecitata dal presidente Follini con una lettera a lei diretta del 26

alle sue decisioni. Ciò che è certo è che, per ragioni politiche e regolamentari, che attengono alla dignità di questo Parlamento, lei deve farci votare queste mozioni.

lei ha risposto parzialmente alle questioni che ho posto, non solo ieri, ma soprattutto stamattina. Innanzitutto perché la mozione che abbiamo presentato, se fosse stata ritenuta impropria, la Presidenza l'avrebbe dovuta dichiarare inammissibile. In realtà, non ho mai proposto di mettere ai voti una richiesta che non poteva comunque essere messa ai voti perché nell'ordine logico deliberato dalla maggioranza la decisione sulla preclusione totale o parziale delle mozioni spetta a lei in questa fase, e non prima, cioè al momento del voto sulle dimissioni. Detto ciò, credo che, richiamando anche una sua dichiarazione di ieri, vi sia l'esigenza che talvolta la sostanza prevalga sulla forma. In questo caso, la sostanza coincide con la forma perché al netto della mia mozione (di cui lei può disporre come ritiene, anche se non condivido e contesto la sua decisione) comunque le mozioni dei colleghi di maggioranza e di opposizione del Partito Democratico e del Popolo della Libertà non sono, e non possono considerarsi, precluse totalmente perché contengono due proposte: l'una, che riguarda la decadenza del senatore Di Girolamo, che è preclusa o assorbita - come dice lei - dal voto; l'altra, che riguarda la revoca dell'ordine del giorno De Gregorio che resta in piedi. Rispetto a quest'ultima, avevo chiesto anche oggi, signor Presidente, qualora - e non ne comprenderei le ragioni - la maggioranza e l'opposizione non intendessero chiarire che quello non è un precedente, come lei ha fatto nella lettera al Presidente della Giunta (e credo che questo sarebbe un elemento di serenità), se lo può dichiarare lei a nome dell'Aula. A me sta bene: non è infatti il problema formale del voto, ma piuttosto il problema istituzionale, la rimozione di un precedente nefasto, che non serve ai lavori della Giunta. L'altra questione che ho posto stamattina - alla quale lei, signor Presidente, non ha risposto - riguarda il modo in cui noi nella Giunta delle elezioni dobbiamo procedere per il subentro del signor Fantetti al senatore Di Girolamo. Ciò in quanto il parere espresso dall'allora presidente del Senato Marini nel 2006 riguarda solo la procedura di subentro per chi è stato eletto al Parlamento nazionale nelle circoscrizioni nazionali, per cui si pone il problema dei limiti dei poteri della Giunta delle elezioni. Stamattina, infatti, ho sollevato la questione, che è su tutti i giornali e che credo comunque debba investire anche la responsabilità istituzionale di ciascuno di noi: mi riferisco al fatto che il collega che dovrebbe subentrare può anche darsi che abbia alcuni problemi in ordine ai requisiti di eleggibilità, dal momento che sembra essere dipendente di un Ministero, precisamente del Ministero delle politiche comunitarie, da tempo. Il requisito per il mantenimento di questo rapporto d'impiego è la residenza in Italia e la residenza in Italia non consente l'elezione

che succede nell'ordine; viceversa, se - come è, se non vi è un'estensione del parere del presidente Marini - dovesse andare a fare una verifica in ordine ai requisiti sul subentro, è chiaro che tutto questo avrebbe bisogno di un altro tipo di indicazione. Noi dobbiamo quindi andare avanti.

ha votato, sia in Commissione che in Aula. Cosa facciamo una volta che lo dichiariamo decaduto? Facciamo la rivisitazione di tutte le votazioni per vedere se c'è il principio di resistenza?

a un accertamento di mancanza dei requisiti per la candidatura e per l'elezione (requisiti che sono fatti risalire al momento della proclamazione, ossia al 2008) rispetto alle dimissioni, i cui effetti maturano da oggi. Il titolo di senatore

candidata. Attraverso questa procedura noi impediamo invece di rimuovere tutte le conseguenze giuridiche connesse all'elezione a senatore, che non possono ovviamente essere vanificate e annullate dalle semplici dimissioni che operano da oggi. Ciò che si è già consolidato come diritti, in base al titolo e alla funzione ricoperta di rappresentante e di componente di quest'Aula, rimane acquisito. che la decadenza impedisca che si possano consolidare i diritti collegati alla proclamazione a senatore e, poiché la Giunta sostiene

Sulla tematica della Giunta delle elezioni e l'invito a me rivolto in ordine al subentrante,

Per quanto riguarda il dibattito, colleghi, non ho molto da aggiungere, nel senso che la Conferenza dei Capigruppo di ieri ha seguito un percorso che è stato confermato dal voto dell'Aula. in proposito quanto ho letto ieri in Aula sull'esito della Conferenza dei Capigruppo: «Qualora non dovessero essere accolte le dimissioni predette, si passerà all'esame delle mozioni concernenti la relazione della Giunta sull'elezione contestata nella circoscrizione Estero e, in caso di approvazione delle mozioni medesime, l'ordine del giorno dell'Assemblea si intenderà immediatamente integrato

tracciato una linea: la preclusione del voto sulle mozioni in presenza di accoglimento delle dimissioni. Non entro nel merito, mi limito a dettare l'esito della Conferenza dei Capigruppo, poi confermato dal dibattito in Aula, alla luce del diniego del voto contrario alle richieste dell'opposizione, che andavano su due percorsi.

poi ho messo ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore D'Alia, nel senso di votare la mozione da lui presentata anche in caso di accoglimento delle dimissioni, la quale ugualmente non è stata della tenuta del calendario dei lavori, approvato - seppur a maggioranza - in Conferenza dei Capigruppo. Non è quindi nei poteri discrezionali della Presidenza integrare oggi l'ordine del giorno: ricordo ai colleghi, anche dell'opposizione, che vi sono altri strumenti per chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno

dopodiché, lei dice che la decisione assunta è stata confermata dal dibattito. Voglio solo ricordarle che, prima in Conferenza dei Capigruppo, in maniera assolutamente esplicita e franca (e credo che i colleghi lo ricordino),

come abbiamo dimostrato durante due giorni di dibattito, dal voto sulle dimissioni e che era quella della revoca dell'ordine del giorno del senatore De Gregorio. Infine, osservo che ci sono molti, molti modi per condurre il dibattito e dirigere il Senato, e ce ne è uno che noi decisamente non apprezziamo: far finta che le parole non siano mai state pronunciate e che le richieste non siano mai state avanzate.

Signor Presidente, vorrei ricordare, mi rivolgo alla Presidenza, ma faccio riferimento a quanto testé detto dalla senatrice Finocchiaro, che l'ordine del giorno De Gregorio, che ciascuno è libero di condividere o non condividere, e a suo tempo è stato libero di votare o non votare,

non voglio polemizzare, e mi astengo quindi dal fare considerazioni. Mi attengo ai fatti e le faccio una proposta. I fatti sono questi: il collega Malan è primo firmatario di una mozione che chiede la revoca di questo fantomatico ordine del giorno;

di revocare l'ordine del giorno del senatore De Gregorio. Solo questo: è un capoverso comune a tutte e tre le mozioni, di maggioranza e di opposizione. Se lo si vuole trasformare e riformulare,

La conclusione cui approdano le tre mozioni è identica: non dobbiamo aggiungere significati politici, diamo un significato giuridico a ciò che stiamo facendo, e limitiamoci a questo, peraltro nello spirito, signor Presidente, di quella saggia lettera che lei ha inviato e che noi, come Giunta, non abbiamo potuto soppesare adeguatamente proprio perché ci trovavamo dinanzi all'ordine del giorno. giorno. Nello spirito di ciò che lei ci sollecitò a fare, condiviso da tutti i Gruppi, stiamo compiendo un atto meramente giuridico. Nessun altro commento è opportuno che si faccia: si rimuova quel richiamo al giudicato e quindi quell'ordine del giorno che vincola le nostre decisioni da adottare nel rispetto dell'articolo 66 della Costituzione, a prescindere dagli accertamenti di altra autorità.